Presidente, in queste ore stanno arrivando dal Venezuela notizie impressionanti... Sono notizie impressionanti per tutto il mondo; forse per uno che ha fatto un ululato in quest'Aula non sono impressionanti, ma è uno su più di trecento. Per noi sono impressionanti*. (Applausi

portati. Vorrei che il Senato, che è stata la prima voce che si è levata per solidarizzare con il Parlamento e con il popolo venezuelano, mandasse un messaggio chiaro: dell'incolumità fisica di questi due esponenti e *leader* venezuelani è, a pieno titolo, responsabile il presidente Maduro, per tutto quello che potrà succedere nelle prossime ore. Le famiglie, infatti, ci chiedono di lanciare questo appello a difesa dei diritti delle persone e della loro incolumità fisica. Ieri il presidente Gentiloni Silveri e il nostro ministro degli affari esteri Alfano hanno usato parole chiare, limpide e trasparenti. Hanno parlato di deriva totalitaria e dittatoriale, con votazioni imposte al popolo di un'Assemblea costituente che in alcun modo l'Europa e l'Italia riconoscono.

a solidarizzare, ancora una volta, con il Parlamento venezuelano, con gli italiani, connazionali, angosciati in queste ore, e con il popolo che sta in piazza contro una dittatura narcomilitare, è un atto che nobilita il Parlamento e la nostra sensibilità internazionale.

del rapimento di suo padre, avvenuto solo poche ore fa. Credo sia un atto dignitoso del nostro Parlamento far sentire la voce di ogni Gruppo politico,

così da consentire che non ci sia uno Stato che si senta padrone della loro vita. *(PD)*. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo del Partito Democratico, in assoluta sintonia e assonanza con quanto il presidente Casini ha

avendo la consapevolezza, che ci veniva dai *report* di quel Paese, dagli oppositori e dai parlamentari in fuga, che eravamo di fronte a una deriva che avrebbe portato alla guerra civile e alla fine della democrazia e alla dittatura. Eravamo di fronte a una deriva davvero molto pericolosa. Il primo atto che il presidente Maduro ha adottato - lo voglio ricordare al Parlamento della Repubblica - è stato togliere l'immunità ai parlamentari,

Adesso si è compiuto un atto finale. Attenzione, perché questi atti portano progressivamente, magari sulla base di ragioni economiche e di una delle più grandi crisi economiche che il Paese ha attraversato (non solo per responsabilità dei Governi che

il popolo, ma anche gli stessi concetti di libertà e democrazia. In questo senso, siamo in assoluta sintonia con il presidente Casini e con le parole che ha pronunciato sul Venezuela, terra che a noi sta a cuore per i nostri connazionali, per quel popolo

Signor Presidente, concordiamo anche noi del Gruppo per le Autonomie - Partito socialista - MAIE con le parole del presidente Casini e degli altri colleghi che sono già intervenuti. tuttavia, non richiamare i fatti di questa notte e non ricordare a quest'Assemblea e a tutti noi che queste sono cose che abbiamo già visto: le abbiamo già viste in giro per il mondo, ma le abbiamo viste anche nel nostro Paese (è soltanto di qualche mese fa l'anniversario del rapimento di Giacomo Matteotti e della sua successiva uccisione). Concordo con le parole del presidente Casini nel ritenere, nel caso accadesse qualcosa a questi due esponenti politici dell'opposizione venezuelana, come primo

battaglia popolare venezuelana per la democrazia. Non capisco come certi pezzi della sinistra italiana non si associno a questa battaglia di affermazione di democrazia e di principi di libertà: non ci può essere interesse di bottega, non ci può essere solidarietà con altri Stati che in questo momento in Venezuela giocano una partita magari discutibile da parte di Gruppi politici italiani. Per quanto mi riguarda, il mio futuro sarà ancora di impegno politico in questo Parlamento, ma sarà difficile condividere con loro prospettive politiche che in questo momento li fanno dividere da un impegno solidale di questo Senato.

su questo tema così importante e delicato, che riguarda anche nostri connazionali che hanno portato cultura, lavoro, onestà, dignità e tanti esempi di cosa significa essere italiani in quel Paese, così lontano ma nello stesso tempo così vicino. Non c'è dubbio che l'impostazione, prima di Chavez ed oggi di Maduro, che è nata da una protesta senza proposta, ha portato quel Paese, signor Presidente, la ventesima economia al mondo, dotato di straordinaria ricchezza e di grandi opportunità sotto tutti gli aspetti, in una situazione devastata e devastante. Non può continuare così. Credo sia giusto e doveroso che il Senato ed il Governo si impegnino con concretezza nel mandare un messaggio forte e chiaro di vicinanza ai nostri connazionali, ma, nello stesso tempo, anche al presidente Maduro che così non si può andare avanti. *(Applausi

noi abbiamo sottolineato come la situazione stesse degenerando per quanto riguardava gli aspetti di democrazia, di libertà e di sicurezza in quel Paese. È troppo tempo che anche cittadini di origine italiana sono stati ammazzati, nel silenzio assordante di tante istituzioni, mentre protestavano per difendere i loro diritti e la loro libertà. Oggi noi siamo solidali con quanto detto dal presidente Casini, condividiamo a pieno questo appello e speriamo che la comunità internazionale non sia assente rispetto a ciò che sta avvenendo in Venezuela e che anche il Governo italiano faccia sentire forte la sua voce

Signor Presidente, è per me del tutto naturale associarmi alle dichiarazioni del presidente Casini e dei colleghi che mi hanno preceduto,

Peraltro, come parlamentari italiani, abbiamo il vantaggio che in quest'Aula sieda il collega Orellana, che in Venezuela ha vissuto a lungo e che giornalmente ci fornisce notizie e ci presenta dati sullo sviluppo della situazione. Qual è il dato veramente impressionante? È il fatto che Maduro sta imponendo non semplicemente un monopolio d'autorità, che espropria il Parlamento delle sue legittime funzioni di rappresentante della volontà popolare ma, per così dire, un monopolio politico che estromette gli avversari e i contendenti dall'arena e dalla scena politica. Oltre al fatto che la storia di questi giorni è costellata di incidenti, di uccisioni, di sparatorie, di interventi che umiliano la dignità umana e la dignità dei singoli soggetti. soggetti. Dobbiamo anche denunciare un fatto. È in corso, e molti parlamentari ne sono stati vittime, una sorta di *mail bombing* da parte di nostri connazionali, i quali si ostinano caparbiamente a negare la realtà dei fatti,

e trarre appunto auspici perché il Paese possa vedere rapidamente il ripristino della regola democratica nella sua pienezza.

La tragedia venezuelana è iniziata già prima di Maduro, ma equilibri cosiddetti demagogici o ideologici impedivano di parlarne. L'intervista rilasciata questa mattina dice una cosa allucinante: l'Assemblea costituente farsa, da lui fatta eleggere con tutti i mezzi militari e polizieschi a disposizione, servirebbe - lui lo dichiara con una semplicità unica - a punire e a fare arrestare tutti i parlamentari. Il Parlamento non deve esserci, il Parlamento deve tacere; c'è solo la sua voce. Un popolo ridotto alla fame da tempo, per scelte che alcuni anni fa erano anche orgogliose, ma poi rivelatesi disastrose, negando ogni democrazia. Noi, però, parliamo sempre

Questo è il dato reale. Se poi la democrazia deve essere una battaglia di facciata e la si difende solo se ci fa comodo, non è una battaglia ma è una farsa e le farse non sono accettabili. In Venezuela è in atto una tragedia. Dobbiamo muoverci e anche noi dobbiamo contribuire, insieme all'Europa e a tutti gli altri, a sanzioni ulteriormente pesanti, anche se allucinanti (a un popolo martoriato si impongono altre sanzioni), con la speranza che questo signore vada a casa vada a casa da solo, senza ulteriori traumi per un Paese e ulteriori vittime. Egli, infatti, è solo un volgare dittatore della peggiore specie. Ma di questi personaggi in giro per il mondo ce ne sono tanti. E se crediamo in una democrazia vera dobbiamo denunciare tutto questo. Con quanto silenzio

Per chi abusa di tutti e apre e chiude le porte del proprio Paese in termini di ricatto? Questo è il dato reale. Quindi, in generale si abbia coraggio: l'Italia sia un Paese in cui la democrazia trionfa e che vuole che trionfi ovunque. Questa è la vera battaglia. Piena solidarietà al Venezuela e piena solidarietà a tutti i Paesi che vivono quel tipo di condizioni! Presidente, io e i colleghi del mio Gruppo parlamentare non abbiamo mai avuto, nel corso di questi mesi, da quando è cominciata la crisi in Venezuela, alcuna esitazione ad applaudire le parole di tutti quelli che hanno provato a mettere in campo uno sforzo per la ricerca della pace e di una soluzione condivisa, non erano personaggi secondari del dibattito pubblico e politico che ha attraversato il mondo. Il primo a dire cose di questo genere, cioè a chiedere che tutti gli attori in campo nella drammatica vicenda venezuelana facessero un passo indietro, è stato il Papa, con parole solenni, dichiarate molti mesi fa Il secondo è stato l'ex*premier* spagnolo Zapatero, che è stato, come sappiamo, per molte settimane in quel Paese. Anche lui ha cercato, nei limiti del possibile, in una situazione che andava degenerando giorno dopo giorno, di mettere in campo sforzi diplomatici e un tentativo di portare il Paese fuori dalle secche di una possibile guerra civile.

omette di parlare delle cose esattamente come stanno - che ho più dubbi ad applaudire quando la vicenda del Venezuela viene rappresentata come se ci fosse da una parte un Governo dittatoriale e dall'altra parte, invece, una opposizione fatta di gentiluomini che si batte per la democrazia. Io non ho alcuna remora a dire ad alta voce che contesto e non condivido il comportamento del Governo Maduro. Lo considero sbagliato e considero sbagliate, ovviamente, le repressioni di tutte le forme di dissenso democratiche credo che, anche rispetto alle speranze che nel corso degli anni passati erano state suscitate dai primi anni della rivoluzione bolivariana e dal chavismo, questi comportamenti siano molto sbagliati e dannosi. Ma francamente questa idea, che davvero sento soltanto nel Parlamento italiano perché in altri Paesi del mondo vi è un po' meno sufficienza su questo e un po' più di approfondimento,

L'opposizione venezuelana è certamente rappresentata dai giovani che manifestano nelle piazze, associazioni di uomini e donne che si battono per la democrazia e per i diritti umani. A loro va tutta la nostra vicinanza. Ma l'opposizione venezuelana di questi mesi è stata anche e soprattutto il ritorno di elementi conosciuti in tutto il mondo come riconosciuti golpisti fascisti. anni e nel corso degli anni passati è stata addestrata alle scuole paramilitari della CIA in America Latina *(Applausi dal Gruppo Misto)* e che è stata complice delle peggiori dittature sudamericane nel corso degli ultimi trent'anni.

degli errori e dei limiti del Governo Maduro, ma francamente questa idea davvero tutta italiana (che, insisto, non trova riscontri in alcun'altra parte del mondo) di considerare

che Papa Francesco sia un riferimento di tutti in quest'Aula, non può succedere che qualche volta le sue parole si ascoltino e qualche volta invece, quando danno fastidio, si ascoltino di meno. Io Papa Francesco lo ascolto sempre e quando lui ci invita a fare attenzione, a non contribuire a far sprofondare quel Paese nella guerra civile, a trovare soluzioni e a non immaginare una dinamica di parte che possa essere, quella sì,

sulla questione venezuelana. Da parte nostra non si ci sarà alcuna difesa dell'indifendibile e metteremo in campo tutte le forme di distanza che occorrono verso politiche repressive che non hanno niente a che vedere con quello che pensiamo noi, quelle di Maduro e di una parte molto significativa della sua classe dirigente. Ma insisto: non si può far diventare tutti i soggetti dell'opposizione venezuelana, compresi i golpisti fascisti, i nuovi campioni della democrazia; su questo, mi dispiace, ma il Gruppo di Sinistra Italiana esprime una distanza

Non c'è problema e non mi sento offeso per questo. Volevo però garantire ai colleghi che avevo chiesto la parola per tempo. Signor Presidente, vorrei esprimere, a nome del Gruppo, la solidarietà all'opposizione venezuelana e la condivisione delle parole espresse dal presidente Casini. Vorrei anche chiarire che oggi non stiamo parlando di errori e limiti del Governo Maduro, ma stiamo parlando di dichiarazioni e atti insopportabili e in aperto contrasto con qualsiasi regola democratica. che le opposizioni sono diversificate, ma quando si colpisce l'opposizione, si colpiscono tutte le opposizioni e non è consentito fare distinzioni. Così come non è un caso che, quando questo accade, avviene sempre attraverso un'azione che indebolisce innanzitutto le prerogative dei Parlamenti. È accaduto anche questa volta. ciò ci dovrebbe portare, colleghi, a due riflessioni: innanzitutto ad avere molta attenzione per il parlamentarismo, le sue tradizioni e le sue prerogative, a condannare quegli atti di antiparlamentarismo che sono molto facili da identificare. Noto che anche nel dibattito corrente c'è una grande attenzione e una condanna più o meno quotidiana per il cosiddetto populismo, che è una categoria assolutamente incerta e indefinita, laddove invece c'è molta più tolleranza per gli attacchi al Parlamento, sia quando questi vengono perpetrati a casa nostra, sia quando accade in casa d'altri, laddove invece l'attacco al Parlamento, rispetto a ipotetici populismi, è molto più facile da individuare e anche da contrastare. Credo che su questo abbia ragione il collega Tarquinio: dovremmo essere assolutamente rigidi in questa condanna e dovremmo manifestarla sempre. È evidente che ogni situazione è diversa dall'altra, ma quando c'è un attacco al Parlamento c'è un indebolimento della democrazia. Questo è avvenuto ieri in Turchia, oggi in Venezuela. Sarebbe bene che i liberi Parlamenti se ne accorgessero sempre,

la capacità di respingere gli attacchi dei suoi nemici diventa evidentemente più flebile. Signor Presidente, d'altra parte questa cosa si spiega conoscendo la storia e il suo andamento. Lo vorrei dire al collega Buemi. Cambiano le sigle dei partiti, molto spesso cambiano le bandiere e i simboli, cambiano i riti, ma è molto più difficile che cambino le mentalità. È per questo che in una discussione come quella di oggi è possibile rintracciare continuità con un passato che apparentemente è passato ma che invece, se si considerano le mentalità, è un passato che non

Signor Presidente, ci troviamo a riesaminare il testo del disegno di legge sulla concorrenza perché, come è noto, la Camera - lei lo ha ricordato - ha apportato cinque modifiche. La prima riguarda l'abrogazione del comma 01 dell'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, modifica introdotta al Senato, relativo alle polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia contenute nel comma 25. La Camera dei deputati ha abrogato la parte, introdotta proprio dal Senato, che prevedeva che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potessero essere rinnovate tacitamente, riportando l'articolo al testo originario.

dal senatore Girotto, su cui a lungo avevamo dibattuto. Esso prevedeva che gli operatori di telefonia avessero l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione una serie di dati identificativi del soggetto committente e, inoltre, che non si potessero più offrire servizi in abbonamento senza il previo consenso espresso e documentato. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva evidenziato, già al Senato,

Ciò sarebbe stato in contrasto con le direttive europee sulla *privacy* e così la Camera ha abrogato tale disposizione. La terza modifica riguarda il comma 60, *ex* articolo 29, relativo alla cessazione del regime di maggior tutela per l'energia elettrica, sul quale si soffermerà più diffusamente di me ilsenatore Tomaselli. La quarta modifica, relativa al comma 153, *ex* articolo 57, riguarda l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche all'interno di strutture sanitarie. È una norma che precisa che le prestazioni odontoiatriche devono essere svolte solo e unicamente dai soggetti abilitati secondo legge, ma forse alla Camera si è andati oltre le migliori intenzioni, tant'è che la 10a Commissione del Senato ha approvato un ordine del giorno chiarificatore; altrimenti sarebbe stata incerta la presenza di odontoiatri in strutture pubbliche. Queste quattro modifiche sono state approvate in Commissione alla Camera; l'Assemblea della Camera ha poi modificato il comma 117, *ex* articolo 44, relativo alla razionalizzazione della rete dei carburanti si sono realizzati degli equivoci. Nel corso dell'esame al Senato il comma era stato modificato prevedendo la bonifica del sito solo in caso di accertata contaminazione; la Camera ha modificato il testo inserendo le parole «in ogni caso» e questa nuova definizione porta a una formulazione che suscita qualche dubbio interpretativo, tanto per cambiare.

Autorevoli rappresentanti della maggioranza alla Camera avevano accolto il disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Senato il 3 maggio con agguerrite dichiarazioni circa il fatto che il Gruppo di maggioranza assoluta alla Camera avrebbe approvato il provvedimento solo in presenza di forti modificazioni.

il comma 60 sulla maggior tutela non è una modesta correzione. In Senato nel mese di aprile di quest'anno abbiamo suggerito un rapido passaggio in 10a Commissione per apportare quelle modifiche e quei miglioramenti che il lasso di tempo intercorrente tra l'agosto 2016 (quando la 10a Commissione

per attualizzare il disegno di legge. Il Governo ha invece insistito per un rapido passaggio in Assemblea con il voto di fiducia. Pensavo che anche la Camera a quel punto avesse preceduto con il voto di fiducia, invece in quel ramo del Parlamento si è aperta una fase emendativa che ha richiesto questo quarto passaggio. Non mi sembra che le modifiche apportate, comunque, abbiano migliorato il testo. Ognuno di noi ha un'idea della concorrenza e non può che essere così, perché se è sbagliato un mercato chiuso, è anche sbagliato un mercato senza regole e senza limiti. Ognuno di noi si è fatto un'idea di questo disegno di legge e soprattutto del perché abbia impiegato così tanto tempo per uscire dalle Aule parlamentari. Sul ritardo accumulato se ne sono dette tante, si sono espresse valutazioni critiche spesso infarcite di luoghi comuni, di banalità e di pregiudizi, ad esempio quello sul peso delle *lobby* come motivazione di questo ritardo. È una sciocchezza, come è folkloristico l'elenco dei lobbisti e addirittura l'individuazione di una saletta-gabbia dove rinchiuderli, come è avvenuto alla Camera dei deputati, come se non esistessero i telefoni e i contatti personali al di fuori del Parlamento. Il disegno di legge in discussione è rimasto fermo per tanto tempo per le esigenze della politica, non per le *lobby*. Vorrei aggiungere che i settori toccati dal testo in discussione hanno una oggettiva complessità. Occorre favorire i consumatori, senza però dissestare il sistema delle imprese e degli altri operatori economici. Occorre tagliare le rendite, ma non il profitto. Occorre recuperare errori che si sono sedimentati nel tempo, ad esempio le parafarmacie, senza abbattere speranze ed energie imprenditoriali. Non sono temi facili e non possono sempre essere risolti con un tocco di bacchetta magica. Non so se quella previsione legislativa, che doveva essere uno stimolo e un pungolo a governare i processi, cioè quella di realizzare ogni anno una legge sulla concorrenza, sia una previsione da rivedere. Ma è indubbio che, in materia di liberalizzazioni e di concorrenza praticata e non terrorizzata, ci sono campi ancora da arare in profondità. In questo disegno di legge abbiamo affrontato ad esempio i temi della RC auto e delle energie. Ma quanto c'è da fare circa l'azione monopolistica delle società a forte partecipazione di capitale pubblico, che si interessano ad esempio di acqua e le cui tariffe medie sono aumentate in un anno, anzi in dieci anni, del 90 per cento? Se prendiamo l'anno di riferimento del *referendum* sull'acqua, cioè il 2011, notiamo che da allora ad oggi le tariffe dell'acqua sono aumentate del 43 incrementi superiori a qualunque altro servizio di tipo pubblico e superiori di gran lunga all'inflazione sui prezzi al consumo, che si attesta intorno al 14 per cento. Ho parlato dell'acqua perché è un tema di attualità. Ma le tariffe sui rifiuti sono cresciute in dieci anni del 52 per cento e i trasporti del 30 per cento. Ci sono poi temi sui quali il dibattito e la diversità di opinioni tra di noi, ma anche il dubbio circa le ricadute positive sui consumatori sono un arricchimento e non un pregiudizio o una difesa di interessi lobbistici. Ad esempio, la norma sul tacito rinnovo in campo assicurativo, che ci viene riproposta dalla Camera (quindi la Camera ha bocciato la proposta del Senato), farà risparmiare il consumatore o l'assicurato? Io penso di no; io penso che le tariffe RC auto siano diminuite, certo, per la diminuzione delle truffe e degli indennizzi, ma forse anche perché non c'è più il tacito rinnovo, che impone all'impresa assicuratrice ogni anno di riconquistare il cliente. la norma sul *telemarketing*, modificata anche questa dalla Camera, ripristinando il testo precedente e vanificando l'azione del Senato. Noi l'abbiamo introdotta accettando un emendamento del Gruppo Movimento per aiutare il consumatore e per difenderlo dall'invadenza e talvolta dall'aggressività del venditore, per tutelare il suo consenso. La Camera e anche il garante, legittimamente, ritengono invece che l'effetto sarebbe opposto e controproducente. la norma sulla nullità delle clausole contrattuali degli albergatori che utilizzano piattaforme digitali, senza neppure aver accolto l'introduzione della clausola cautelativa. Questa è davvero una norma tre una norma tre volte vincente, cioè vincono i consumatori, vincono gli albergatori e vince lo Stato italiano? Io penso di no. Io penso che per gli albergatori si potrebbe prevedere invece un aumento, una tassa d'ingresso quando debbono accedere ai portali, per lo Stato si potrebbe prevedere una procedura di infrazione, mentre il cliente probabilmente pagherebbe le stanze come prima. Ma io non dispongo della verità, non ho la sfera di cristallo. Penso che si debbano rispettare le regole, soprattutto se contratte tra privati, e che, tanto per non generare equivoci, gli *over the top* digitali debbano pagare le tasse in Italia, bloccando evasione ed elusione. E allora perché dico tutto questo? Lo dico non per rinfocolare una polemica, ma all'opposto. Penso che, sulla concorrenza e su temi così delicati e difficili da discernere, le convinzioni diverse e le valutazioni critiche ci stanno tutte e da tutte le parti, ma è sul complesso del provvedimento che occorre esprimere il giudizio, perché non esiste perché non esiste un disegno di legge sulla concorrenza perfetto per tutti i palati. Due scienziati dell'economia e della concorrenza hanno scritto sul «Corriere della sera» che questo disegno di legge va approvato «anche solo per non darla vinta alle *lobby*». È inutile negarlo: qualche *lobby* ha ottenuto ciò che voleva o ha ridotto i danni (è inevitabile), ma questo disegno di legge va approvato non per quello che dicono gli scienziati dell'economia, bensì perché rappresenta un ulteriore passo in avanti della concorrenza nel nostro Paese. Non sarà una legge epocale, ma certamente rappresenta un'evoluzione moderna in molti settori dell'attività economica. Il saldo tra le cose buone, quelle che si potevano fare meglio e le forzature è certamente più che positivo. Sarà un provvedimento incisivo e riformatore. Apportare nuove modifiche a uno o a tutti i cinque commi introdotti dalla Camera in terza lettura potrebbe comprometterne il traguardo: sarebbe la caduta del ciclista in dirittura d'arrivo. Per questo noi relatori abbiamo chiesto, insieme al Governo e ai commissari della 10a Commissione, il ritiro o altrimenti la bocciatura di tutti gli emendamenti, alcuni dei quali certamente apprezzabili. I consumatori, le categorie professionali, il mondo produttivo e dei servizi, le istituzioni europee ed internazionali hanno bisogno non di rinvii, ma di certezze. Abbiamo consumato in abbondanza il tempo a nostra disposizione. D'altra parte, se Governo e Parlamento avessero preso alla lettera le norme esistenti della legge sulla concorrenza, oggi avremmo oggi avremmo dovuto fare il terzo provvedimento sulla concorrenza. E approvando oggi questo provvedimento, non arretriamo, non stiamo fermi: facciamo non uno, ma due passi in avanti sul piano dell'ammodernamento e della competitività del nostro Paese.

La discussione sulla questione di fiducia, per la quale è stata ripartita un'ora e 30 minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi, si svolgerà, fino alla sua conclusione, nella seduta pomeridiana odierna, con inizio alla ore 16, dopo l'esame del bilancio interno del Senato. Le dichiarazioni di voto avranno inizio domani, in seduta unica senza previsione di orario di chiusura, a partire dalle ore 9. Seguirà quindi la chiama. L'ordine del giorno di domani prevede inoltre - ove richiesto dal prescritto numero dì senatori - la discussione su atti di indirizzo relativi alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali e l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2016. La seduta antimeridiana di oggi proseguirà con la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza sul disegno di legge in materia di abolizione dei vitalizi. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 12 settembre, alle ore 17, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. La Conferenza dei Capigruppo è convocata, sempre martedì 12 settembre, alle ore 15.30. L'attività ordinaria delle Commissioni riprenderà a partire da lunedì 4 settembre. Le Commissioni sono comunque autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.

nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. Ha la parola il senatore Cappelletti per illustrare la richiesta.

la storia di questo provvedimento per meglio comprenderne la portata e soprattutto per capire come siamo arrivati a formulare la richiesta odierna di calendarizzazione d'urgenza del provvedimento che è già stato approvato alla Camera. Appena entrati in Parlamento noi del Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto due cose: abolire i vitalizi degli ex parlamentari, applicando anche a loro il ricalcolo contributivo, e abolire la pensione privilegiata degli attuali parlamentari, anch'essa un vitalizio mascherato che manda in pensione gli onorevoli a sessantacinque anni dopo solo quattro anni, sei mesi e un giorno in Parlamento. In sostanza, abbiamo chiesto che anche i parlamentari prendano la pensione esattamente con le stesse regole applicate a tutti gli altri italiani. A settembre del 2013 il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per mettere un tetto ai vitalizi e alle pensioni d'oro e ricalcolare la quota contributiva. PD e maggioranza hanno votato no. Nel 2014, durante la discussione sul bilancio della Camera e del Senato, il Movimento 5 Stelle ha presentato un ordine del giorno che prevedeva un tetto massimo di 5.000 euro lordi ai vitalizi. Partito Democratico e la maggioranza hanno votato no. Il 20 maggio 2015 il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento alla riforma costituzionale che intendeva abolire i vitalizi in Costituzione. Il Partito Democratico e la maggioranza hanno votato no. Il 9 luglio 2015 il PD, evidentemente sotto pressione, tramite Matteo Renzi ha presentato la cosiddetta legge Richetti, ma l'ha presentata in televisione perché giace da anni in un cassetto, anche se veniva utilizzata spesso dallo stesso Renzi durante le apparizioni televisive per dire che il Partito Democratico è per il superamento, per l'abrogazione. Arriviamo Arriviamo a noi: il 2 aprile 2017 il Movimento 5 Stelle ha presentato in Ufficio di Presidenza altri due ordini del giorno, uno che applica la legge Fornero ai parlamentari in carica e l'altro che ricalca la stessa legge Richetti. Sul primo, ancora una volta, il PD vota no perché ha sostenuto che serviva una legge ordinaria. Benissimo, allora calendarizziamola questa legge ordinaria e votiamola, cosa che è stata fatta anche e forse soprattutto grazie alla spinta mediatica di trasmissioni televisive molto seguite nel Paese che hanno destato l'attenzione importante dell'opinione pubblica su questo argomento. La verità dunque, signori, è che il PD si è sempre opposto. Nella recentissima votazione alla Camera sembrava di assistere ad un funerale. Io capisco che per voi rinunciare ad un diritto che somiglia veramente ad un privilegio di tipo medievale è una cosa innaturale, però l'avete comunque votata alla Camera, forse nella malcelata speranza che il disegno di legge possa essere insabbiato analogamente ad altre dozzine di emendamenti. Ora, io capisco bene che la democrazia è anche e soprattutto una questione di numeri ma la trasparenza è un importante ingrediente della democrazia. Chiedo quindi, con il voto sulla dichiarazione di urgenza, di rendere palese a tutti i cittadini italiani se siete favorevoli o no al mantenimento di questo privilegio di stampo medioevale, o, almeno una volta, di essere coerenti con quanto avete dichiarato, e cioè di essere favorevoli a un suo veloce superamento. Delle due l'una e, se non è abbastanza chiaro il concetto, torno a ribadirlo con le vostre parole. Vengo a ribadire le motivazioni a favore della dichiarazione di urgenza, citando le parole usate da voi, dai vostri parlamentari, commentando il voto favorevole alla Camera sul provvedimento.

Camera ha detto: «Non possiamo più permettere disparità di trattamento così forti e ingiustificate. Tutti meritano di andare in pensione, ma nessuno può pretendere di ricevere più di quanto ha versato.

«Bisogna votare sì perché il punto è capire che la disuguaglianza è un male vero nella nostra società, che va affrontato con misure concrete tutt'altro che demagogiche»: siete sempre voi. Benissimo. Ma forse più chiaro di tutti è Matteo Renzi: «Grazie a Matteo Richetti e ai deputati del PD, orgoglioso del vostro lavoro sui vitalizi». «La legge Fornero, se vale, vale per tutti. Le stesse regole per i cittadini e per i politici». Presidente, dichiarandosi orgoglioso del lavoro dei parlamentari del PD sui vitalizi, a quale lavoro faceva riferimento Matteo Renzi? A quello che ha portato, tra mille ostacoli, il disegno di legge a essere approvato alla Camera o a quello di insabbiamento che è ora in corso al Senato che potrebbe avere inizio proprio oggi con la bocciatura di questa dichiarazione di urgenza? Valutatelo voi. Per il Paese e per i cittadini italiani tutti i vitalizi vanno abrogati subito. Il Movimento 5 Stelle non ha dubbi e voterà favorevolmente alla dichiarazione di urgenza. Gli altri Gruppi risponderanno del loro voto alle loro coscienze e sopratutto ai cittadini.

il nostro Gruppo voterà contro la dichiarazione di urgenza, innanzitutto per una ragione di metodo: questo disegno di legge

e va approfondito. Se questo vale per un ufficio studi, a maggior ragione vale per ogni singolo parlamentare su una questione che evidentemente non è secondaria. C'è poi una ragione di merito che ci porta a prendere questa decisione: noi siamo fermamente convinti che un principio contenuto in questa norma, cioè quello della retroattività, sia manifestamente incostituzionale. Non è una convinzione soltanto nostra, signor Presidente, ma è una convinzione che è stata espressa a chiare lettere da esimi costituzionalisti, ex presidenti della Corte Costituzionale di destra, di centro e di sinistra. Evidentemente c'è una ragione. Se questo è vero noi rischiamo un cinico *spot* elettorale sulla pelle dei cittadini italiani. Non costa niente votare un provvedimento come questo, se si è certi che la Corte costituzionale interverrà, come ha fatto in passato, per abrogarlo dopo pochi mesi. Se invece ciò non dovesse avvenire, signor Presidente, passerebbe un principio

lo stato di diritto, ma ancor più mette in forse le certezze economiche di quel ceto medio che è stato colpito duramente dalla crisi. Vorrei che tutti i colleghi riprendessero le dichiarazioni del presidente Boeri che dice di volere riconsiderare le pensioni cosiddette d'oro a partire da 3.500 euro. Signor Presidente, una pensione di 3.500 euro non è d'oro

si rapporta difficilmente nei confronti dei suoi cittadini. Noi questo vorremmo evitarlo. Non c'è alcun altro motivo, se non ragioni di equità,

decidere, come Senato, una tassa di scopo ben elaborata che si raccordi ai princìpi costituzionali, o un contributo di solidarietà, perché in un momento così difficile dai parlamentari venga un segno chiaro e inequivocabile, noi saremmo i primi ad aderire a questa proposta e, anzi, ci faremo parte in causa, perché questa possa essere la soluzione per cui

conosciuto approfonditamente e il testo stesso fa sì che siano parecchi i punti di dubbia interpretazione. È pertanto difficile esprimersi compiutamente su un testo concepito in siffatto modo.

I casi sono due: il provvedimento sarà considerato incostituzionale dalla Corte costituzionale oppure non lo sarà, perché sarà ritenuto compatibile con la Costituzione. Se la Corte costituzionale lo dichiarerà incostituzionale, come moltissimi esperti di diritto costituzionale hanno ampiamente previsto,

azioni che riguardano questioni assai più ampie e meno giustificate di una pensione. La parola vitalizio è un inutile eufemismo. Si chiamano pensioni vitalizie perché così fu deciso da Camera e Senato nell'immediato dopoguerra.

L'altra ipotesi è che invece poi in qualche modo le norme contenute nel presente disegno di legge, una volta approvate definitivamente, siano

Le pensioni dei parlamentari sono certamente più alte della media delle pensioni degli italiani, perché il reddito annuale di un parlamentare è mediamente più alto di quello dei cittadini; vi sono però molti cittadini che percepiscono

migliaia di eccezioni, hanno la loro pensione calcolata sulla base del sistema contributivo a partire dal 2011, quando entrò in vigore la legge Fornero in tutti i suoi vari aspetti, e con il calcolo retributivo per quanto riguarda

un assegno di pensione, ma anche a coloro che già lo percepiscono, comprese le vedove e i vedovi che, come tutti i vedovi e le vedove di pensionati italiani, hanno una quota di reversibilità,

pressoché d'obbligo - e forse questo a qualcuno piace - passare a un ricalcolo contributivo retroattivo per tutte le pensioni di tutti gli italiani, e anche di coloro che oggi

contenere le spese, porre rimedio ad alcuni parametri ingiustificati, che infatti sono stati tutti soppressi, salvo quanto riguarda il passato.

passare all'esame del provvedimento in titolo senza l'inutile dichiarazione che serve a fare un titolino o un titolone, a seconda dell'interesse dei giornali a occultare altre notizie assai più importanti.

penso all'incompatibilità della pensione del parlamentare con cariche che ancora ricopre anche al di fuori del Parlamento - in precedenza non era così - nonché al limite ai cumuli e così via.

Signor Presidente, condivido quanto ha anticipato il senatore

come hanno detto i miei colleghi - da esperti costituzionalisti. A me è balenata soltanto una prima considerazione: il collega del parla di uguaglianza di tutti i cittadini, e quindi anche dei parlamentari, sotto il profilo previdenziale. Allora chiedo ai chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle: non ritenete voi, nel momento in cui viene approvata una norma con effetti retroattivi,

sapendo di avere il sistema contributivo negli anni passati, ha ritenuto di riscattare ad esempio gli anni della laurea, del servizio militare e quant'altro, per organizzare a a suo vantaggio il proprio sistema previdenziale? Oggi, il deputato che si vede retroattivamente applicare il sistema contributivo quale possibilità ha di fare la stessa cosa che hanno fatto tutti i cittadini che avevano quel sistema contributivo? Un provvedimento di tal genere dovrebbe allora essere accompagnato da una riapertura dei termini anche per i deputati che oggi si vedono retroattivamente applicare un sistema contributivo. Anche Anche a loro deve essere data la possibilità di usufruire di quelle agevolazioni di cui tutti i cittadini, con quel sistema, hanno goduto. A questo non ci avete pensato. Avete immaginato soltanto di cavalcare l'onda

una distinzione tra me e chi svolge un'attività diversa dalla mia. Ma chi è che percorreva e denunciava quasi ogni domenica questi fatti? Chi, per condurre una una manifestazione canora nazionale nel nostro Paese, ha guadagnato, dai soldi degli italiani, 650.000 euro per cinque giorni di lavoro?

poi in televisione va a criticare il vitalizio dei deputati. Signori, a prescindere dal merito, che non mancherà di essere da me attenzionato anche sotto il profilo squisitamente tecnico,

voler urgentemente licenziare un provvedimento di tal genere soltanto per dare una possibilità di marchette elettorali a determinate forze politiche.

una volta, dai giudici della Corte suprema di cassazione e della Corte costituzionale che è un provvedimento sbagliato. Per questa ragione, noi diciamo no, un no deciso e convinto. Con coraggio diciamo no oggi al voto della dichiarazione d'urgenza. Ci riserveremo poi, nel merito dell'esame del provvedimento, di verificare e valutare se davvero si pongono tutti sullo stesso piano, deputati e cittadini, perché io su questo punto sono d'accordo con il Movimento 5 Stelle: devono essere tutti i uguali i cittadini italiani, ma lo devono essere per davvero. attenzione, perché il provvedimento che è arrivato qui dalla Camera a me pare non rispetti il principio di uguaglianza. Ovviamente approfondirò il tema

- ma lo voteremo soltanto quando ci saremo convinti della bontà del provvedimento sotto il profilo della sua costituzionalità, del merito e dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte al sistema previdenziale. previdenziale. Per queste ragioni, allo stato, diciamo no alla dichiarazione d'urgenza. Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE non vede alcuna necessità per un'abbreviazione dei tempi

ci stiamo occupando di temi molto delicati, considerato soprattutto che la proposta di legge in esame incide pesantemente sui diritti acquisiti degli ex parlamentari. Si tratta quindi non di insabbiare la questione, ma di valutarla attentamente, di fare una legge fatta bene, per non finire poi davanti alla Corte costituzionale di compiere un grande pasticcio. Ricordo ai colleghi che un'analoga questione si è posta in Regione Trentino-Alto Adige, dove il Consiglio regionale

il nuovo regime in contrasto con i criteri dettati dalla Corte costituzionale in materia. Per noi si tratta anche di una questione di civiltà giuridica e crediamo che i principi costituzionali debbano valere per tutti i cittadini, anche per i parlamentari e per gli ex parlamentari. Per questo motivo voteremo no alla richiesta di urgenza presentata dal Movimento 5 Stelle.

avanti da molti mesi a questa parte. Signor Presidente, io ho difeso la dignità di questo Senato da chi voleva abolirlo con il *referendum* costituzionale in maniera improvvida. E l'ho difesa assieme alle colleghe e ai colleghi del mio Gruppo quando ho sostenuto la necessità, ancora oggi, di una centralità del bicameralismo. Troverei, quindi, davvero contraddittorio se oggi il Senato dovesse svolgere

ma farò le barricate se qualcuno pensa di poterlo utilizzare come un grimaldello per attaccare le normali pensioni degli italiani. Se qualcuno, cioè,

per il Paese e anche per la credibilità della sua classe dirigente. Signor Presidente, in questo dibattito ho ascoltato vari interventi che hanno affrontato il merito del disegno di legge sui vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Tuttavia, oggi noi siamo chiamati a discutere e a votare non nel merito, bensì sulla richiesta di adottare una procedura d'urgenza per un provvedimento di cui tutti - lo dimostra il dibattito che abbiamo ascoltato - riconoscono l'importanza e la delicatezza. La richiesta d'urgenza viene dai senatori del Movimento 5 Stelle che - desidero sottolinearlo, in quanto è l'unica occasione che ho per farlo - è l'unico Gruppo che stamattina non ha preso la parola per condannare il regime

ritardare - come stiamo facendo - l'inizio del dibattito finale su un provvedimento di grande rilievo, come quello sulla concorrenza, così atteso...

Perché questa inversione di priorità da provvedimenti che interessano i cittadini italiani a un dibattito su procedure di palazzo? Io credo che nella risposta a queste domande ci sia la principale ragione per cui le senatrici e i senatori del Partito Democratico respingeranno la richiesta di urgenza... Il Movimento 5 Stelle continua a praticare una politica parlamentare che - è evidente - punta non su ciò che è più urgente per risolvere i problemi dell'Italia,

ha un obiettivo chiaro: vogliono apparire agli occhi dell'opinione pubblica italiana come i campioni dell'antipolitica, dell'antipartitismo e come i rappresentanti delle forze antisistema. Questo è l'obiettivo.

Presidente, se le cose stanno così, è bene che ci mettiamo d'accordo sui principi e sui modi che dovranno regolare la nostra discussione sulle pensioni dei parlamentari, cominciando proprio dal fatto che dobbiamo cessare di chiamare vitalizi quello che dal 2012 è stato trasformato dal Parlamento in un regolare sistema pensionistico contributivo. Le senatrici e i senatori del PD vogliono esaminare con rispetto ed attenzione un provvedimento così rilevante che ci arriva dalla Camera con il voto dei deputati del Partito Democratico e con la prima firma nostra, e non certo quella del Movimento 5 Stelle. Il Senato non deve dilungare la discussione e non lo farà, ma non deve troncarla artificialmente. Al Senato, in questa legislatura, il Partito Democratico non ha mai - e dico mai - praticato tecniche ostruzionistiche che, invece, sono usate continuamente proprio da chi oggi chiede l'urgenza. E non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo certamente ora. Anzi, vigileremo perché in Commissione e in Aula i lavori procedano con regolarità. Come tutti i provvedimenti, vogliamo esaminare anche questo con lo scrupolo necessario, studiandone il contenuto e gli effetti, valutandone l'impatto sul sistema parlamentare e i risvolti di costituzionalità, che non sono certamente aspetti secondari e che la Commissione ha il dovere primario di valutare con la necessaria attenzione. Ricordava adesso il senatore De Cristofaro che il *referendum* del 4 dicembre ha detto con chiarezza che gli italiani vogliono conservare il sistema bicamerale paritario. Chi, come me, ha votato sì alla riforma deve essere il primo a essere molto rigoroso nel rispettare la volontà degli elettori. Ma anche chi, come il Movimento 5 Stelle, ha votato no ha l'obbligo morale di rispettare la sostanza e non solo la propaganda del significato e dello spirito del bicameralismo. Una Camera, quella dei deputati, davanti a un provvedimento difficile, ha discusso per anni; l'altra Camera, il Senato, viene invece incitata a votare in tempi brevissimi, immediatamente, già il 1° settembre - come ho sentito dire dall'opposizione e questo non corrisponde al modello di bicameralismo che il *referendum* ha confermato. *(Applausi È significativo che il Movimento 5 Stelle, che nelle piazze ha fatto del no al *referendum* la sua bandiera, oggi, con una richiesta d'urgenza così intempestiva e così sterile, voglia imporre una procedura che ridurrebbe il lavoro del Senato a quello di un mero passacarte, impegnato più nel rispetto... *(Commenti dei senatori Senatore Petrocelli, la richiamo all'ordine: non interrompa. Chiedete la parola quando volete, ma non interrompete. Prego, Senato che vorreste impegnato nel rispetto di una velocità imposta e non nello studio del provvedimento. Ho terminato, signor Presidente, ma una considerazione politica devo svolgere in chiusura. C'è molto cammino da fare perché chi predica una democrazia nella quale un *clic* conta più della volontà dei parlamentari possa apprezzare la maturità di una democrazia parlamentare rappresentativa e il senso positivo delle sue procedure.

Presidente, debbo dire che veramente non si accorgono che stanno usando dei metodi da regime. *(Applausi

parla di democrazia diretta noi dobbiamo intendere che la vuole diretta da altri centri di potere. Vuole che in Parlamento Signor Presidente, il disegno di legge sulle pensioni dei parlamentari farà allora in Senato il suo corso regolare, rigoroso, senza alcun rallentamento e senza alcun trucco, né per intralciarne la trattazione né per modificarne il cammino. I senatori del Partito Democratico hanno un'unica richiesta da fare su questo provvedimento: che venga esaminato con serietà, con scrupolo, attenzione e senza demagogia. E che la discussione democratica del Senato sia pure vivace ma resti sempre all'interno di quel comportamento civile che questa mattina non ho visto e che è l'unico modo conosciuto per costruire dei buoni provvedimenti. *(**Applausi

Sull'ordine dei lavori e per fatto personale,

intervengo per denunciare la gravissima situazione ambientale di Aprilia. *In primis* vorrei segnalare i numerosi esposti presentati da diversi cittadini, singoli e associati, supportati da una documentazione imponente su problemi relativi a violazioni ambientali rimaste ad oggi completamente ignorate. Io stessa ho sollevato con un atto ispettivo la situazione di un terreno agricolo in Via Nettunense 102 all'interno del quale era stata rilevata una illecita attività di stoccaggio e commercio di prodotti chimici per l'industria e l'agricoltura, nonché rifiuti speciali pericolosi e tossici di vario tipo. Ho chiesto al ministro Galletti urgenti iniziative di competenza affinché sia previsto un percorso finalizzato a garantire la rimozione dei rifiuti

Alcuni giorni dopo la mia interrogazione, è stata sequestrata nel territorio di Aprilia, in località Tufetto - una zona sottoposta a vincolo idrologico - una enorme discarica abusiva. cui sorgente si trova *in loco* non viene imbottigliata, ma fino a pochi giorni fa è stata liberamente usata dai cittadini della zona. L'operazione Dark Side ha portato a sedici le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sei divieti di dimora, più sequestri di società, fabbricati, terreni, automezzi, conti bancari e contanti per 15 milioni Si ipotizzano reati che vanno dall'associazione a delinquere al traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. a parte il sito di via Nettunense e a parte quello della cava, ci sono tanti altri episodi per i quali a si può ravvedere la necessità di chiedere un commissariamento. Ci sono discariche abusive da bonificare dalla fine degli anni Ottanta.

normativa Seveso non viene rispettata, non è stata mai fatta una sola esercitazione, e non sono reperibili i piani di emergenza. In definitiva ad Aprilia (ma non solo lì ovviamente) il lassismo e l'incuranza su aspetti così fondamentali per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia ambientale

che sono stati rapiti nel corso di questa notte. Ringrazio chi ha condannato questa deriva autoritaria e ringrazio anche chi ha chiesto un dibattito aperto e approfondito sul Venezuela, come il collega De Cristofaro, perché sono certo che lo ha fatto in perfetta buona fede. Ricordo però che domenica è avvenuto un fatto gravissimo: un'esigua minoranza di venezuelani è andata al voto e ha eletto un gruppo di 545 persone per costituire una cosiddetta Costituente, caratterizzata dalla presenza di rappresentanti delle corporazioni con divieto di affiliazioni partitiche. Per l'ennesima volta è stato esautorato il Parlamento, eletto con suffragio universale un anno e mezzo fa. Al suo posto ora c'è una Costituente illegittimamente indetta (ricordo che sarebbe dovuta essere preceduta da un *referendum*) e invece ciò non è avvenuto. Dalle nostre comode poltrone possiamo disquisire ora su questa o quella dichiarazione di esponenti dell'opposizione, su questo quell'orientamento politico, ma resta il fatto indubitabile e incontrovertibile della fine della democrazia in Venezuela. Lo dico il cuore spezzato, perché il dolore è molto forte per questa situazione: si sta tornando agli anni bui della dittatura degli anni Cinquanta. Questo deve essere chiaro a tutti. L'Italia deve prendere una posizione netta

Presidente, non volevo che passasse la giornata senza ricordare in questa Assemblea la figura di Nicola Cipolla, che è morto a Si spegne un'altra personalità e protagonista del lungo e travagliato cammino della democrazia italiana e dell'altrettanto travagliato e tragico percorso della politica siciliana. Nicola Cipolla è nato nella città di Pirandello, ad Agrigento, dove passò la sua gioventù. Si trasferì con la famiglia a Palermo, dove al Liceo classico «Umberto I» ebbe compagni di classe della personalità e del calibro di Napoleone Colajanni, Enzo Sellerio, Nino Sorgi. Fu anche per lui l'occasione per entrare dentro la temperie culturale del suo tempo, ma anche per conoscere e apprezzare la cultura marxista. Con la fine del fascismo si aprì la stagione nuova della speranza e Cipolla aderì al PSI e fu tra i fondatori del Fronte del lavoro. Oggi riposa proprio nella camera ardente della CGIL di Palermo, che allora, nel 1944, contribuì a riaprire insieme con Cesare Cessa. Nel 1946 Cipolla ingaggia una battaglia

il sindaco di Palermo fu reintegrato nel Partito Socialista e fatto eleggere nella Costituente. Cipolla decise di rompere con il suo partito e aderì al Partito Comunista, guidato in Sicilia da un'altra spiccata e carismatica personalità, Girolamo Li Causi. Il suo percorso si avvia attraverso il lavoro sindacale nel cuore della struttura sociale del Mezzogiorno, l'agricoltura, dove si forgiavano le giovani classi dirigenti. Basti pensare su tutto allo stesso Pio La Torre. Nel 1947 venne eletto segretario responsabile della prestigiosa Federterra. Iniziò così l'epopea delle lotte contadine con l'occupazione delle terre incolte dei grandi e sterminati feudi e per la riforma agraria, la mamma di tutte le riforme. Tra il 1949 e 1950, insieme a Pio La Torre, vive le lotte per la terra a Corleone, avendo alle spalle la memoria di Bernardino Verro, che all'inizio del Novecento fu protagonista del primo ciclo delle lotte contadine attraverso quel vasto e ricco movimento dei Fasci siciliani. Sempre a Corleone conobbe personalità del calibro di Placido Rizzotto, avendo anche di fronte a sé nei mesi di quel tempo le cosiddette prime stragi di Stato con lo sterminio dei migliori *leader* e dirigenti per mano della mafia, degli agrari reazionari, delle istituzioni colluse, sino a giungere alla strage di Portella della Ginestra, quella che viene ormai comunemente definita la prima strage di Stato.

Nel 1963 arriva in questa Aula del Senato nelle file del Partito Comunista, candidato nel collegio di Sciacca, una provincia molto progressista in quel tempo. Viene confermato senatore nel 1968 e dal 1° luglio del 1963 fino al 14 novembre del 1967 è segretario del Gruppo del Partito Comunista, un ruolo che impone molta severità e capacità sia organizzativa che politica. Nel 1972, alla sua terza legislatura, viene confermato al Senato nell'altro collegio progressista di Ragusa. Dal 1972 al 1976 è membro della rappresentanza italiana al Parlamento europeo. Nel 1981 fonda il Centro studi di politica economica in Sicilia Si dedica così alle tematiche del movimento della pace e, di recente, a quelle attuali dello sviluppo sostenibile, una bella memoria per un tempo odierno arso di cultura progettuale e di sane passioni politiche.

la situazione allo stato della discussione e quello che sarebbe successo in assenza di provvedimenti seri sull'azienda. Ad un anno da quella discussione e dall'approvazione di quell'ordine oggi ritorna prepotentemente la richiesta dell'amministrazione capitolina e del sindaco Raggi di un aiuto economico da parte del Governo.

«A valutare la possibilità di collocare temporaneamente la partecipazione dell'ATAC all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, affidando contestualmente a una struttura tecnica scelta *ad hoc* il compito del risanamento industriale e patrimoniale dell'azienda». signor Presidente, perché, ritenendo e continuando a ritenere che l'ATAC sia un patrimonio pubblico del Paese e che non è un'azienda di trasporto pubblico come le altre, in quanto serve la Capitale d'Italia e quindi non solo i cittadini romani,